di diversa articolazione in Commissione nel Senato. Il punto di riferimento della nostra interpellanza sono i cosiddetti LEA, quei livelli essenziali di assistenza che vennero introdotti nel Servizio sanitario nazionale con la riforma del 1992. Erano allora definiti una sorta di indicazione di prestazioni indispensabili e fondamentali, che dovevano essere assicurate in tutto il territorio nazionale, in quanto - era questo il senso della riforma - si diceva che essi costituissero, più che una priorità, un qualcosa di irrinunciabile per i cittadini, con le risorse assegnate dal Fondo sanitario nazionale. Cosa è accaduto nell'arco di questi vent'anni? Che, di fronte ai crescenti disavanzi delle Aziende sanitarie locali, la considerazione economica ha preso inevitabilmente il sopravvento, e un maggior rilievo sulle esigenze del sistema di tutela della salute e su quella previsione di carattere nazionale fissata dalla legge. Così si

come prestazioni essenziali - e si è cercato di garantire, a livello nazionale, che ne fosse assicurata copertura con le risorse assegnate, imputando poi, nei fatti, alle Aziende sanitarie locali eventuali costi superiori praticati *in loco*. più o meno imminente, del cosiddetto federalismo fiscale - di qui la sollecitazione di un senatore, come il sottoscritto, che non è né un esperto, né si occupa di sanità, a differenza dei colleghi Calabrò e Gustavino e Gustavino - ha inevitabilmente preso piede una sorta di predeterminazione nazionale dei bisogni da assicurare in sede locale, trattandosi di materia trasferita alle competenze regionali, garantita in questa competenza dalla Costituzione, nonché ovviamente l'inevitabile resistenza alla predeterminazione di costi standard slegati dai modelli organizzativi realizzati in sede locale, che è venuta sommandosi alla severità della crisi economica complessiva che ha investito il nostro Paese. Le ricadute più pesanti in materia di tutela della salute hanno allora fatto sì che di fatto - lasciando stare le enunciazioni i cosiddetti LEA, i livelli essenziali di assistenza, vengono riferiti e legati a singole prestazioni. Di qui una sorta di ripiegamento su quei tre macrolivelli essenziali di assistenza obbligatoria in tutto il sistema sanitario nazionale e, anzi, condizione perché si possa parlare di sistema sanitario nazionale, riferiti all'obbligo di garantire ovunque

Nell'ambito della questione che ha investito la nostra sensibilità, riferita ai cittadini sopravvissuti ad esperienze di tumore - e ricordo che parliamo di circa 2 milioni e mezzo di persone noi avevamo pensato, e di qui il ricorso allo strumento dell'interpellanza, di suggerire all'Esecutivo,

una nuova formulazione del titolo dedicato alle neoplasie, superando quella genericità sulla quale si è imbattuto finora

interpellanza - il Governo può ipotizzare una sorta di quarto macrolivello, riferito proprio a quella assistenza molteplice e multivariata che segue il superamento di di patologie gravissime, come i tumori, per renderla obbligatoria in tutti i contesti regionali. riferimento perlomeno a quella necessità di assistenza domiciliare integrata, che non può essere rimessa alle condizioni a noi sembra che questo quarto macrolivello meriti una sorta di priorità nelle risorse del Fondo sanitario, abbia una sua autonomia rispetto al macrolivello dell'assistenza ospedaliera

su quei livelli minimi di assistenza multivariata *post* acuzie nelle patologie tumorali, da contemplare, perlomeno come linee guida, alle Regioni, e quindi di sottrarre alla previsione dell'esercizio dell'autonomia regionale. Tutto ciò, a prescindere da quello che è il giudizio su come questa o quella Regione o, più in generale, l'istituzione regionale, ha esercitato le linee fissate dal legislatore nel 1992. Con questo spirito, dei senatori Gustavino e Calabrò, abbiamo ritenuto che questo problema fosse strettamente legato,

la salute*. In via preliminare si osserva che la definizione dei costi standard utilizzata per la costruzione del fabbisogno standard, come descritto nel capo IV del decreto legislativo attuativo della delega contenuta nella legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale, è diversa dal concetto teorico di costo standard. In termini teorici, il costo standard corrisponde - difatti - con il costo di produzione di un bene o un servizio in condizioni di efficienza ottimali, valutando come non ottimali i costi della produzione che man mano si discostano dal costo standard. Proporsi l'obiettivo di valutare, per trarne uno standard, i costi effettivamente registrati nelle varie realtà osservate, presuppone che i prodotti (*output*) per essere confrontabili sotto il profilo dei loro costi di produzione (*input*) siano omogenei in tutte le loro caratteristiche. Ciò comporta che una adeguata definizione dei costi standard presuppone che nelle singole Regioni siano stati implementati sistemi di controllo e di contabilità analitica e colmata ogni eventuale carenza di dati sui flussi di produzione e dei sistemi gestionali. Nonostante il fatto che il sistema di contabilità del Servizio sanitario nazionale sia notevolmente evoluto e standardizzato rispetto ad altri settori della pubblica amministrazione altrettanto caratterizzati da un forte decentramento, tali carenze, in molte realtà regionali, ancora oggi sono rilevanti e determinano, in alcune realtà, disallineamenti tra dati gestionali e registrazioni contabili, inficiando così la determinazione e l'applicazione del costo standard, per cui non è detto che i costi (*input*) siano correttamente attributi allo specifico *output* che hanno generato e siano facilmente reperibili. D'altra parte, un costo medio non permette di risalire alle singole funzioni cui si riferisce, ma alla prestazione sommariamente intesa. Di ciò si è tenuto conto, quando si è ancorata la prima determinazione dei costi standard ai tre macroindicatori, citati anche dal senatore Compagna, della prevenzione, della della prevenzione, della assistenza distrettuale e dell'assistenza ospedaliera, in modo da minimizzare errori dì stima che sarebbero inevitabili se si fossero scelti indicatori di maggiore dettaglio. Si fa presente, peraltro, che i servizi sanitari vengono prodotti (o garantiti) in base a caratteristiche e modalità che sono peculiari delle singole Regioni, come interazione tra una specifica domanda sanitaria e caratteristiche organizzative della struttura di offerta; le Regioni, infatti, godono - come si sa - di ampia autonomia nella determinazione del modello organizzativo assistenziale e si differenziano quindi notevolmente tra loro sotto questo profilo. Valutati i costi, nella definizione del fabbisogno finanziario delle singole Regioni occorre tenere conto, oltre che delle caratteristiche della popolazione, anche delle caratteristiche del territorio (contesto socio-economico e morfologia del territorio) e delle connesse peculiarità dei servizi offerti. Nel rispetto delle valutazioni che abbiamo appena reso e nel merito della questione sollevata, questo Ministero fa presente che l'attuale accezione di costo standard da utilizzarsi, in applicazione del predetto decreto legislativo, a decorrere dal 2013 per parametrare il riparto delle risorse finanziane del Servizio sanitario nazionale noto, dalla cornice finanziaria in coerenza con il quadro macroeconomico - comporta che esso sia computato a livello aggregato per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza prima riferiti, e non sia calcolato, pertanto, per singola prestazione, ma per gruppi di prestazioni associabili ai Va evidenziato, inoltre, che la determinazione dei costi standard è da considerarsi come un processo. Il tutto richiede che, nelle singole Regioni e nelle singole aziende sanitarie siano implementati sistemi di controllo e di contabilità analitica, sia colmata ogni eventuale carenza di dati sui flussi di produzione e sui sistemi gestionali, come abbiamo detto. Allorché sarà disponibile una periodicità sistematica di ricezione dei dati relativi a tali indicatori, potrà essere rimodulata con maggiore dettaglio la definizione dei costi standard per singole aree prestazionali. pertanto, questo Ministero può rassicurare gli onorevoli interpellanti sull'adozione di iniziative atte a garantire progressivi miglioramenti dei processi informativi, di programmazione e di controllo rispetto all'attuale quadro normativo che è sicuramente perfettibile sulla base delle esigenze via via emergenti. Da ultimo, questo Ministero ritiene fondamentale che per garantire la sostenibilità del sistema occorra accompagnare le misure di determinazione del costo standard con manovre strutturali e di recupero dell'efficienza, soprattutto nelle realtà dove si registrano cospicui disavanzi. Solo in questo modo si potrà ottenere che le risorse messe a disposizione dallo Stato restino vincolate ai fondamentali obiettivi di miglioramento del Servizio sanitario nazionale, individuati congiuntamente dallo Stato e dalle Regioni.

colleghi - che prendere atto con soddisfazione, se non addirittura con gratitudine, della disponibilità mostrata da parte del Ministero della salute.

amministrazione di settore, così prestigiosamente rappresentata dal Sottosegretario per la salute, ma proprio in sede di coordinamento, di rapporti con le Regioni e di coesione territoriale. Siamo rispettosissimi delle istanze regionali,

la nostra sensazione è che si possa anche prevedere qualcosa di più, una forma cioè di predefinizione di livelli essenziali di tutela rispetto a

costituisce da un punto di vista quantitativo un aspetto così importante per il quale è pur vero le differenze tra Regione e Regione, sarebbe certamente lesa la Costituzione, però in quel diritto costituzionale alla salute a me sembra difficile, per chi esce da una neoplasia, non far rientrare esigenze di riabilitazione e di assistenza domiciliare integrate, (abbiamo fatto tanti dibattiti anche in questa Aula sulle terapie del dolore, sulle cure palliative, eccetera). Quindi, rispetto alla condizione dei malati oncologici, prendiamo atto volentieri e con gratitudine della disponibilità del del Ministero della salute di quelle che sono le sue prerogative. Ci permettiamo però, nella sede più politica di rapporti con le Regioni e di coesione territoriale (senza fare di queste occasioni un seminario di diritto costituzionale sui limiti e gli ambiti delle potestà regionali), di segnalare come i dati e i termini dei rapporti sulla condizione assistenziale dei malati oncologici, del resto forniti proprio dal Dicastero del sottosegretario Roccella, ci portano insistere nella speranza (senza nulla ledere del regionalismo da potenziare, del federalismo fiscale e di tutto quello che si vuole) i problemi da noi posti possano valere sempre di più in questa prospettiva di Italia federale, che può essere a diverse velocità nella standardizzazione, ma non può giudicare, fuori dell'ambito e dei limiti della politica nazionale, la condizione dei malati di tumore.

Signor Presidente, il Ministero della salute avverte in modo sempre più forte la necessità di strategie vaccinali omogenee e comuni non solo per garantire ai cittadini un uniforme diritto alla prevenzione vaccinale, ma anche perché soltanto comuni strategie possono evitare il rischio che l'ecologia microbica si differenzi tra le diverse aree geografiche del Paese, tanto da rischiare di ridurre l'impatto di contrasto che le vaccinazioni vorrebbero contenere. La legge costituzionale n. 3 del 2001, recante «Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione» (articolo 117), prevede che lo Stato formuli i principi fondamentali in materia di strategie vaccinali, ma non intervenga sulle modalità di attuazione di principi ed obiettivi, perché ciò rientra nella competenza esclusiva delle Regioni. Il Piano nazionale vaccini 2005-2007, adattandosi alla nuova realtà aperta dalla modifica del Titolo V, con un importante tentativo di coordinamento tra le diverse istanze delle Regioni e le necessità complessive del Paese, forniva indicazioni generali per i vaccini per i quali non fosse già previsto un programma esteso di immunizzazione a livello nazionale. Tale Piano, pur nel rispetto dell'autonomia regionale prevista, si proponeva di mantenere un coordinamento delle strategie vaccinali, con la possibilità di offrire una apertura all'introduzione di nuovi vaccini nel Paese, con la gradualità e la programmazione necessaria. Al suo interno, e per mezzo della sua applicazione, veniva disegnata una strategia innovativa per la politica vaccinale del Paese: l'ottimizzazione dell'impegno vaccinale nell'offerta attiva e l'adeguamento dei servizi e della costruzione di un idoneo ed efficiente sistema informativo vaccinale, a partire dalle anagrafi vaccinali fino alla implementazione progressiva delle nuove vaccinazioni. Di fatto, però, riguardo alle coperture vaccinali la situazione non è completamente soddisfacente, In tale contesto si riconferma la necessità di elaborare una strategia condivisa da tutte le Regioni nel rispetto della loro legittima autonomia, il più possibile in armonia con le politiche europee. Sulla base di questi elementi, l'apposito gruppo di lavoro istituito in seno al Consiglio superiore di sanità ha predisposto una bozza di Piano nazionale vaccinazioni per il 2010. Esso si prospetta come strumento di supporto tecnico-scientifico alla Conferenza Stato-Regioni e come guida alla pianificazione delle strategie di sanità pubblica per la promozione della salute. La finalità è quella di garantire un uso ottimale dello strumento vaccinale nella prevenzione delle malattie, una base di riferimento affinché le Regioni possano garantire uniformemente il diritto alla prevenzione vaccinale. La bozza del nuovo Piano prevede la definizione del processo decisionale e dei criteri *evidence* *based* per l'introduzione di nuovi vaccini nel calendario nazionale. Infatti, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha pubblicato nel 2005 un documento che rappresenta un punto di riferimento per i Governi in merito alle decisioni da prendere sull'introduzione di nuovi vaccini. Nelle linee guida dell'OMS vengono illustrati gli elementi chiave che devono essere considerati nel processo decisionale. Tali elementi sono suddivisi in due importanti aree di valutazione: le problematiche di politica vaccinale e le questioni di carattere programmatico. dunque, predisposta una bozza di calendario per l'infanzia che prevede l'offerta attiva e gratuita delle cosiddette vaccinazioni obbligatorie (vaccinazioni che nel corso del tempo sono state rese obbligatorie per legge come l'antidifterica, l'antipolimielitica, l'antitetanica e così via) e raccomandate (contro pertosse, morbillo, parotite, rosolia, infezioni da haemophilus influenzae b-Hib). Questo secondo gruppo include le vaccinazioni fortemente raccomandate, cioè ugualmente utili ed importanti rispetto a quelle obbligatorie, ma che non sono state imposte per legge, in quanto introdotte in un secondo momento, quando parlare di obbligatorietà era anacronistico, considerato il nuovo e più realistico approccio alle vaccinazioni come necessità e diritto di ciascun bambino di essere protetto dalle malattie prevenibili mediante vaccino. A queste vaccinazioni si è aggiunta, a partire dal 2008, quella anti-HPV, attualmente offerta attivamente e gratuitamente alle ragazze nel corso del dodicesimo anno di vita, in quanto al tempo dell'introduzione venne individuato un finanziamento *ad hoc*. Infine, nella proposta sono state inserite anche le vaccinazioni antipneumococco, antimeningococco C ed antivaricella, che diverse Regioni hanno incluso da tempo nei calendari regionali, prevedendone l'offerta attiva e gratuita per tutti i nuovi nati.

questa è indubbiamente uno strumento essenziale per garantire la corretta conduzione delle attività vaccinali ed assicurare il monitoraggio dell'efficienza dell'attività e il controllo dell'efficacia. Il Ministero della salute è da anni impegnato per la sua implementazione. A tale riguardo, si ricorda che il Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita del 2003 individua, tra le azioni prioritarie, l'attuazione di un sistema di AVI per garantire una corretta conduzione dei programmi vaccinali ed aumentare le coperture; il Piano nazionale vaccini 2005-2007 indicava l'AVI come uno dei cardini del sistema informativo vaccinale, prevedendone l'integrazione con quello sulle malattie infettive e con le anagrafi comunali; il Piano nazionale della prevenzione 2005-2007 individuava tra gli obiettivi da perseguire, nell'area progettuale delle vaccinazioni, il «rendiconto oggettivabile del mantenimento/implementazione dei livelli di copertura vaccinali efficaci per il contenimento delle malattie prevenibili, grazie alla realizzazione dell'anagrafe vaccinale informatizzata»; del Servizio sanitario nazionale», del Ministero della Salute, è stato elaborato il documento «Contenuti informativi minimi per la rilevazione delle prestazioni di vaccinazione», approvato dalla cabina di regia il nuovo Piano nazionale della prevenzione 2010-2012 (adottato con l'intesa Stato-Regioni del 29 aprile 2010) stabilisce che i Piani regionali di prevenzione adottati dalle Regioni prevedano anche la continuità delle attività del Piano nazionale della prevenzione 2005-2007 e successive proroghe, per il completamento degli obiettivi non ancora raggiunti ed il consolidamento e l'estensione di quelli raggiunti. Infine, riguardo all'impegno di questo Ministero per la realizzazione di una campagna di informazione e sensibilizzazione per il sostegno ai programmi vaccinali, è opportuno rilevare che quest'anno l'Italia ha partecipato alla Settimana europea delle vaccinazioni, programmata per l'ultima settimana di aprile, con iniziative previste a livello centrale e regionale. Per una settimana, durante il mese di aprile, nei Paesi di tutta la regione si sono svolte attività per informare e coinvolgere la popolazione ed i professionisti sanitari sul tema delle vaccinazioni e per affrontare le sfide future in tale ambito. Queste attività includono convegni, corsi di formazione, la diffusione di materiale informativo, conferenze stampa e tavole rotonde con i decisori politici. La campagna, incentrata su una comunicazione mirata, contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo primario di raggiungere e mantenere elevate coperture vaccinali nella Regione europea La finalità principale di tali interventi è quella di attirare l'attenzione e aumentare la consapevolezza sull'importanza che ciascun bambino sia protetto dalle malattie prevenibili mediante vaccinazione, che si configura, allo stesso tempo, come un diritto e come un dovere sociale.

Presidente, nel diritto alla salute, è compresa l'offerta vaccinale per patologie prevenibili con la vaccinazione e che si sono dimostrate gravi e invalidanti per i bambini. I pediatri italiani hanno studiato e condiviso un calendario vaccinale sul quale esiste un largo consenso. Sarebbe auspicabile che l'offerta vaccinale anche per i vaccini non obbligatori ma fortemente raccomandati dal mondo pediatrico venisse allargata in modo gratuito ai bambini presenti sul territorio italiano ed in modo uniforme nelle varie Regioni, che oggi applicano disposizioni diverse, come diceva anche la sottosegretario Roccella, rendendo l'offerta vaccinale tipicamente a macchia di leopardo. Nel luglio 2010, la FIMP, la SIP e la SITI, in qualità di maggiori organizzazioni scientifiche in ambito pediatrico, hanno lungamente approfondito il tema delle vaccinazioni e realizzato, attraverso una specifica commissione mista, il nuovo calendario vaccinale. Per tale strumento di prevenzione sanitaria, anche sulla scorta dell'esperienza medico-scientifica e dei dati clinico-epidemiologici forniti dalla rete pediatrica delle tre organizzazioni, si ritiene indispensabile che il calendario vaccinale realizzato dalla FIMP, dalla SIP e dalla SITI sia inserito nei LEA al fine di renderne omogenea l'applicazione su tutto il territorio nazionale. Tale sostegno, peraltro, appare oggi ineludibile, soprattutto dopo l'esperienza vaccinale vissuta a seguito della diffusione del virus H1N1 - come diceva il sottosegretario Roccella - che ha evidenziato come, sulle vaccinazioni, esista un effetto *feedback* negativo. Quando l'impatto della malattia è molto forte, è altrettanto forte il desiderio di vaccinazione per evitare gli effetti della patologia, mentre, mano a mano che la malattia scompare, o non appare nella virulenza prevista, si perde la percezione del rischio e dell'importanza di mantenere vive le strategie di prevenzione. È invece importante proseguire con le vaccinazioni, e non mancano i casi che lo dimostrano. Ad esempio, sono ben noti i principali problemi connessi alla rosolia quando tale infezione è contratta in gravidanza, così come sono altrettanto noti i rischi di dare alla luce un bambino affetto da rosolia congenita, cui sono associate diverse possibili malformazioni. Eppure, la proposta di vaccinazione contro morbillo, parotite e rosolia, anche se non è recente, non ha mai goduto dell'obbligo vaccinale. Ciò ha evidenziato un problema di percezione da parte dei cittadini, problema che è alla base di una copertura vaccinale inferiore agli obiettivi, causata dal fatto che la popolazione considera l'obbligo di vaccinazione come un marcatore di importanza che produce, come ragionamento derivato: «se la legge non la prevede, allora la vaccinazione non è importante». esposto, l'inserimento tra i LEA del calendario vaccinale rappresenta un banco di prova per la sanità pubblica. Innanzitutto, perché le forti differenze regionali ci dicono che l'attività locale, la parte organizzativa, la comunicazione fanno la differenza, e poi perché è la dimostrazione di quanto sia diventata complessa la comunicazione. A lungo gli operatori si sono avvantaggiati della presenza della legge che imponeva l'obbligo della vaccinazione senza investire su comunicazione e informazione. invece, oggi, l'educazione sanitaria, il convincimento degli operatori sanitari medesimi sono indispensabili per garantire coperture vaccinali accettabili. L'idea di introdurre nuove forme di vaccinazione con l'obbligo oggi sembra anacronistica. L'obbligo ha una sua storia, una sua ragione, in un'Italia, quella degli anni Sessanta, estremamente diversificata sul territorio per cultura, condizioni economiche e sociali. In quell'Italia, l'obbligo ha consentito di offrire un servizio su tutto il territorio nazionale, e per giunta in modo gratuito. i tempi sono maturi per fare delle vaccinazioni l'oggetto di una scelta consapevole e responsabile, garantendo omogeneità per uno stesso diritto alla salute a tutti i soggetti in età pediatrica, dalla Sicilia alle Alpi. Morbillo, rosolia e parotite, ad esempio, ci stanno a indicare quanto è difficile farlo, soprattutto senza un adeguato sforzo legislativo.

nazionale vaccinale entri organicamente nei LEA. Questo è l'aspetto fondamentale, perché soltanto facendo entrare il Piano nazionale vaccinale dentro i LEA in modo organico potremo ovviare alle diverse alle diverse condizioni in cui la prevenzione vaccinale avviene nelle varie Regioni e, soprattutto, potremo ovviare anche alle considerazioni che tutte le associazioni pediatriche, indipendentemente dall'orientamento politico politico e culturale, hanno messo in evidenza. Quindi questo è un passaggio molto importante, poiché soltanto l'iscrizione nei LEA può rassicurare l'opinione pubblica italiana, a partire ovviamente soprattutto dalle famiglie.

chiara nella risposta. I livelli essenziali rimandano infatti al piano nazionale di vaccinazione che, una volta passato in Conferenza Stato-Regioni, di fatto, è nei LEA. Forse il passaggio non era molto chiaro. Per quanto indicato nell'interrogazione presentata dalla senatrice Sbarbati, concernente alcune problematiche inerenti la liberalizzazione del servizio idrico integrato, si rappresenta quanto segue. Questo Governo ha attuato il programma con il quale si era presentato agli elettori, anche nella parte concernente la liberalizzazione dei servizi pubblici, ivi incluso il servizio idrico integrato: prima con l'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, poi con il cosiddetto decreto Ronchi e, infine, con la norma inserita nel decreto sviluppo, in corso di conversione, che istituisce l'Agenzia per l'acqua. Detto questo, non è mai stato messo in discussione che l'acqua sia qualcosa di assolutamente speciale, e da questo punto di vista il Governo si riconosce pienamente nella linea seguita nel luglio 2010 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la quale ha come noto sancito che l'accesso all'acqua è un diritto umano fondamentale: «l'accesso a un'acqua potabile pulita e di qualità e a installazioni sanitarie di base è un diritto dell'uomo, indispensabile per il godimento pieno del diritto alla vita». L'acqua, infatti, è - come dice anche il Santo Padre - bene essenziale per la vita dell'essere umano sulla terra. Se questo non è mai stato in discussione, va evidenziato che non da ora le autorità comunitarie mostrano di considerare (si veda il "Libro verde sui servizi di interesse generale" di Bruxelles) il servizio idrico come un "servizio di interesse economico generale". Viene a questo riguardo utilizzata, cioè, l'espressione, adoperata negli articoli 16 e 86, paragrafo 2 del Trattato, che nella prassi comunitaria è considerata riferita a servizi di natura economica che, in virtù di un criterio di interesse generale, gli Stati membri o la Comunità assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico. Sicché, gli statuti comunali nei quali sia riportata la dicitura "il servizio idrico è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica" si pongono in contraddizione non tanto con la normativa italiana, bensì con l'ordinamento comunitario. Quanto all'esistenza di misure di controllo pubbliche tendenti a garantire la buona gestione del servizio da parte dei privati, queste erano rappresentate, sino all'emanazione del decreto sviluppo, essenzialmente dai poteri di stimolo attribuiti alla Commissione nazionale di vigilanza sulle risorse idriche (CONVIRI) nei confronti delle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale le quali, in quanto soggetti affidanti il servizio, sono parte del contratto intercorrente con il gestore privato e si trovano di conseguenza nella condizione di far valere, con gli opportuni strumenti, le eventuali inadempienza del gestore. Quanto ai quesiti più specifici, desidero ricordare anzitutto che, con parere del 19 gennaio 2011, il CONVIRI ha chiarito che il mancato rispetto del contratto di servizio

Inoltre, con riguardo alla richiesta se sia praticabile e legittima da parte delle società di gestione la fatturazione di quote presunte a prescindere dal reale consumo, la risposta non può che essere negativa, giacché, come chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 335 del 2008, la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. Vi è dunque uno stretto rapporto di corrispettività, per effetto del quale, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione.

sono essi i primi che rispondono direttamente alle famiglie e alle loro preoccupazioni ed è importante che il Governo tenga presenti le loro indicazioni. Per quanto attiene alla risposta data dalla sottosegretario Roccella in merito alla interrogazione presentata dalla senatrice Sbarbati e da me,

molte delle risposte date tengono presente ciò che è avvenuto nel frattempo. Vorrei tuttavia sottolineare due preoccupazioni. La prima è che non si consideri sufficientemente l'acqua un bene dell'umanità ed un diritto di ogni singolo uomo.

non in tutte le Regioni questo nesso è stato messo in evidenza in modo giusto, e penso ad esempio alla Sicilia. Vi sono

Come viene detto dalla senatrice Sbarbati e da me, riteniamo che l'acqua debba essere considerata tra i beni di interesse comune dell'umanità, e la risposta da lei data non è del tutto convincente, proprio perché non appare robusto il lavoro del Governo, sia sulla sensibilizzazione dei sindaci per la verifica delle garanzie fideiussorie contenute nel contratto di affidamento sottoscritto con le società di gestione, introducendo la responsabilità del gestore in caso di interruzione del servizio affidatogli, sia su altre questioni e quesiti sollevati

il sito di interesse nazionale di Tito in provincia di Potenza è stato inserito tra gli interventi di interesse nazionale individuati dal programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale elaborato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 426 del 1998. Tale programma è stato adottato con decreto ministeriale n. 468 del 18 settembre 2001, e con successivo decreto ministeriale dell'8 luglio 2002 ne è stato definito il perimetro. L'area ex-Liquichimica si estende per circa 52 ettari. Dal 1969 al 1976 la proprietà era della Chimica meridionale spa, specializzata nella produzione di fertilizzanti; successivamente è stata ceduta alla Liquichimica Meridionale spa, per produzione di concimi chimici e attualmente è di proprietà del Consorzio ASI -Consorzio area sviluppo industriale di Potenza. Così come segnalato dall'interrogante, il sito è interessato dalla presenza di rifiuti di diversa natura, tra i quali amianto, fosfogessi, scorie e polveri derivanti dall'attività siderurgica, materie prime, prodotti e residui di lavorazione derivanti dalla produzione di concimi a base di fosforo. Nelle acque di falda sono stati riscontrati superamenti dei limiti normativi per una serie di parametri. L'anno scorso, in data 29 aprile 2010, in occasione della Conferenza dei servizi decisoria, era stato illustrato lo stato delle attività in essere, riguardanti la bonifica dei materiali contenenti amianto, da cui era risultato che il primo stralcio dei lavori di bonifica era stato già da tempo ultimato e certificato dall'Azienda sanitaria locale n. 2 di Potenza. Inoltre, con riferimento al secondo stralcio, riguardante la bonifica dell'edificio deposito - officina, era risultato che gli interventi di rimozione dei materiali contenenti amianto erano stati ultimati il 30 aprile 2009,

raccolta delle acque meteoriche e delimitazione dell'area interessata con installazione di recinzione, si erano conclusi in data 7 luglio 2009; la rimozione dei serbatoi fuori terra contenenti ammoniaca si era conclusa il 26 gennaio 2009. Per la messa in sicurezza e bonifica delle acque sotterranee e dei terreni dell'area and Liquichimica, la tecnica di bonifica individuata per le acque sotterranee è quella del *Pump & Treat*. Il progetto prevede la creazione di uno sbarramento idraulico, realizzato con pompaggio di acqua di falda ed il successivo trattamento delle acque estratte. L'acqua in uscita dal processo di trattamento potrà essere scaricata nel collettore fognario o nel corpo idrico superficiale. Per la messa in sicurezza permanente e bonifica del bacino gessi, avente ad oggetto i rifiuti (fanghi industriali e fosfogessi) depositati in modo incontrollato nel sito all'interno dell'area ex Liquichimica, è prevista la realizzazione di una serie di vasche impermeabilizzate per rifiuti non pericolosi, ai sensi del decreto legislativo n. Il progetto prevederà anche il recupero funzionale dell'area, con la realizzazione di un piazzale di scambio ferro-gomma nell'ambito più esteso del progetto del raccordo ferroviario di Tito scalo. Conferenza dei servizi decisoria del 29 aprile 2010 ha deliberato: di esprimere parere favorevole alla ipotesi di progetto di messa in sicurezza d'emergenza e bonifica della falda e dei terreni presentata; di prendere atto dell'impegno assunto dal Consorzio ASI nella Conferenza dei servizi istruttoria del 25 marzo 2010 e di trasmettere il relativo progetto definitivo di bonifica della falda e dei terreni subordinatamente al recepimento di alcune prescrizioni formulate dalla medesima Conferenza di servizi di approvare il progetto preliminare di messa in sicurezza permanente con recupero funzionale e reindustrializzazione del "bacino gessi"; di prendere atto dell'impegno assunto dal Consorzio ASI nella Conferenza dei servizi istruttoria del 25 marzo 2010 e di trasmettere il relativo progetto definitivo di messa in sicurezza permanente con recupero funzionale del "bacino gessi" all'interno dell'area ex Liquichimica subordinatamente al recepimento di alcune prescrizioni formulate dalla medesima Conferenza di servizi In sede di Conferenza dei servizi istruttoria del 31 marzo 2011 sono stati esaminati e discussi diversi documenti. Con riferimento al «Rapporto sulle attività svolte per la messa in sicurezza permanente della falda acquifera nel periodo gennaio-settembre 2010», trasmesso da ASI ed acquisito al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 2916 del 31 gennaio 2011, è stato osservato che le attività risultano avviate in data 9 gennaio 2009; esse hanno interessato 20 coppie di piezometri e le acque di falda sono state smaltite come rifiuti. Sono risultati inoltre contaminati 8 coppie di piezometri con i seguenti analiti: ferro, manganese, cadmio, dicloroetilene, tricloroetilene, solfati, fluoruri. Gli emungimenti continueranno nei piezometri risultati contaminati. Con nota del 3 marzo 2011, il Consorzio ha comunicato che la Regione Basilicata in merito al progetto di bonifica della falda e dei terreni e alla messa in sicurezza permanente con recupero funzionale del "bacino gessi", è offerta di valutare la possibilità di adottare soluzioni diverse e alternative rispetto a quelle già proposte ed approvate. In particolare, la Regione ha proposto l'utilizzo di barriere reattive in luogo di quelle idrauliche e, per il "bacino gessi", di utilizzare dati relativi aggiornati provenienti dalla realizzazione della nuova rete piezometrica regionale. La Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente, dopo esame istruttorio e sulla base del parere espresso dall'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) in merito al «Rapporto sulle attività svolte per la messa in sicurezza permanente della falda acquifera nel periodo gennaio-settembre 2010» trasmesso da ASI, ha cosi disposto: che l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente validasse i predetti risultati; che il Consorzio procedesse a pompaggi in continuo; che fosse assicurata una attività di emungimento a copertura del monte-valle idrogeologico; che fossero individuati e analizzati i pozzi scelti con funzione di controllo. In relazione al «Rapporto sulle attività svolte per la rimozione dei rifiuti sparsi presenti all'interno dell'area ex Liquichimica di Tito», trasmesso da ASI, è stato richiesto all'ARPAB di provvedere a verificare quanto dichiarato dal proponente. Con riferimento al «Rapporto conclusivo sulle attività di messa in sicurezza di emergenza», all'ASI è stato richiesto: di fornire, per ciascuno degli interventi di messa in sicurezza di emergenza eseguiti ed indicati nel documento, una relazione dettagliata in merito alle attività svolte, alle eventuali verifiche analitiche eseguite per le varie matrici (terreno, acqua e aria), allegando tabelle di sintesi e rappresentazioni cartografiche utili ai fini della comprensione delle attività svolte e del raggiungimento degli obiettivi di bonifica previsti; di effettuare il collaudo delle pareti e del fondo dello scavo in corrispondenza dei serbatoi di ammoniaca e dei rifiuti sparsi rimossi; di prelevare campioni di *top soil* in corrispondenza delle aree soggette a bonifica di materiali contenenti amianto per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di bonifica anche nel terreno, visto che i due certificati di restituibilità rilasciati dalle autorità competenti a seguito delle operazioni di bonifica dei materiali contenenti amianto si riferiscono alla sola verifica delle fibre di amianto nella matrice aria; di evidenziare, anche mediante carte piezometriche e carte di distribuzione degli inquinanti, sia in senso areale che verticale, se l'installazione della barriera idraulica ha comportato sostanziali variazioni nel deflusso sotterraneo e nelle caratteristiche del plume di contaminazione (estensione, direzione e verso di deflusso); di redigere, in accordo con ARPAB, un piano di monitoraggio *post operam* delle acque (a monte e a valle idrologica della barriera idraulica), dei terreni e dell'aria, che consenta di verificare l'effettiva efficacia nel tempo di ognuno degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza indicati nel documento in esame ed eseguiti; un'attestazione, rilasciata dall'ARPAB, in merito all'esecuzione dell'intervento di rimozione dei serbatoi di ammoniaca, secondo la normativa vigente e in linea con quanto indicato nel relativo progetto, in ottemperanza a quanto già richiesto nelle precedenti conferenze; la presentazione immediata delle nuove alternative progettuali, ovvero l'adozione delle iniziative già discusse ed approvate nella precedente Conferenza di servizi decisoria in merito al progetto di bonifica della falda e dei terreni e al progetto di messa in sicurezza permanente con recupero funzionale del bacino gessi. Attesa la valenza ambientale degli argomenti, infatti, non sono accettabili rinvii nell'adozione effettiva di interventi a tutela della salute e dell'ambiente. All'ARPAB, invece, è stato richiesto di provvedere a verificare quanto dichiarato dal proponente. Il Programma nazionale di bonifica ha stanziato per il sito di Tito le seguenti risorse, da destinare in via prioritaria agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione delle aree pubbliche,

dall'ultimo monitoraggio pervenuto al Dicastero risultano impegnati 3.439.839 euro. A favore della regione Basilicata sono stati trasferiti, fin dal giugno 2003, risorse pari a 166.011 euro, a valere dello stanziamento recato dalla legge 23 marzo 2001, n. 93, articolo 20, per la realizzazione di una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e degli interventi di bonifica urgente. In data 14 ottobre 2010, altresì, la Direzione generale competente del Ministero ha sottoposto alla regione Basilicata l'accordo di programma per la messa in sicurezza d'emergenza e bonifica dell'area industriale di Tito

dove operano almeno 85 imprese e centinaia di lavoratori mentre questo piano, da quel che vediamo e sentiamo, stenta a prendere forma.